Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 1° luglio 2009, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la Regione Campania: Alfonso Andria, Teresa Armato, Raffaele Calabrò, Anna Maria Carloni, Franca Chiaromonte, Luigi Compagna, Barbara Contini, Gennaro Coronella, Diana De Feo, Sergio De Gregorio, Vincenzo De Luca, Aniello Di Nardo, Giuseppe Esposito, Vincenzo Fasano, Giuseppe Follini, Pasquale Giuliano, Maria Fortuna Incostante, Cosimo Izzo, Raffaele Lauro, Adriano Musi, Vincenzo Nespoli, Antonio Paravia, Francesco Pontone, Giacinto Russo, Carlo Sarro, Cosimo Sibilia, Silvio Emilio Sircana, Sergio Vetrella, Pasquale Viespoli e Riccardo Villari.

Bubbico, Bugnano

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 3 del disegno di legge. Onorevoli colleghi, per accordi intervenuti tra i Gruppi parlamentari, le dichiarazioni di voto finale, con ripresa televisiva diretta su RAI Due, avranno inizio alle ore 11,45. Sospendo

noi voteremo contro il provvedimento in esame, e il nostro è un no convinto, sia per il metodo che avete seguito che per il merito della legge. Avete posto la fiducia prima alla Camera e poi al Senato perché preferite, al confronto parlamentare con le opposizioni, la subalternità politica e culturale alla Lega Nord. È proprio vero, dopo le elezioni europee i vostri alleati padani vi fanno sentire sempre più il loro fiato sul collo e dettano l'agenda politica e parlamentare di questo Governo. Avete messo la fiducia non per convenienza ma per paura, la paura di essere di nuovo bocciati a scrutinio segreto da quanti nella maggioranza non condividono alcune norme odiose ed inutili contenute in questo provvedimento. Avete avuto paura del *bis* al Senato dove, in prima lettura, siete andati in minoranza su alcune disposizioni in materia di immigrazione, e avete avuto paura della reazione della Lega. Come si può, allora, votare un provvedimento che dovrebbe servire a migliorare la sicurezza degli italiani e che, viceversa, è frutto di un mero calcolo politico? Un provvedimento espressione di suggestioni, anche stravaganti, che obbediscono alle esigenze della propaganda politica piuttosto che alla reale necessità di sicurezza degli italiani. Noi abbiamo sempre tentato di fare proposte di buon senso per migliorare questa legge. Alcune - poche per la verità - accolte; tante, troppe bocciate per principio, per convenienza e non per convinzione. Nell'arco di un anno questo è il terzo provvedimento che adottate sulla sicurezza: due decreti-legge e questo disegno di legge. Se sulla stessa materia intervenite tre volte in appena dodici mesi significa che la vostra strategia non funziona e che ci sono problemi; significa che avete necessità di alzare sempre di più il livello della propaganda con trovate singolari ed inquietanti come le ronde, il permesso di soggiorno a punti e la cancellazione anagrafica dei bambini stranieri figli di irregolari per coprire la totale inefficacia della vostra azione di Governo. Di questo passo dove arriveremo? Continuate a spendere i soldi dei contribuenti per utilizzare l'Esercito sulle strade. I militari che, per carità, fa piacere vedere passeggiare nei centri storici, costano di più e possono fare meno, molto meno dei poliziotti e dei carabinieri perché da soli non possono né fermare né arrestare nessuno. Perché non utilizzate le stesse risorse per garantire l'ordinario *turnover* delle forze di polizia? Forse perché il vostro ministro della difesa, come ha dichiarato in una delle sue ultime oltre che innumerevoli interviste ed esternazioni, il gerarca La Russa, si è convinto che anche lui ha delle competenze da esercitare sulla sicurezza interna del Paese? Avete imposto le ronde, questa inutile quanto pericolosa scorciatoia che apre la strada alla giustizia "fai da te" e alla costituzione di associazioni con finalità politiche, mediante organizzazioni di carattere militare, espressamente vietate dall'articolo 18 della Costituzione. Sì, colleghi, perché cos'è la Guardia nazionale italiana fascista, con tanto di aquila imperiale sul basco, appena nata e già ribattezzata "ronda nera"? E cosa sono le ronde padane se non associazioni politiche che, in forza di questa legge, esercitano funzioni di pubblica sicurezza e quindi militari?

L'ordine e la sicurezza sono infatti patrimonio esclusivo dei cittadini, di tutti i cittadini attraverso lo Stato e voi, sottraendo competenze allo Stato, le date ai partiti, inaugurando una nuova e pericolosa stagione della giustizia politica italiana. Essa, per definizione, è priva di garanzie e di regole proprio perché si affida alle scelte di una parte contro l'altra. Ed avete la presunzione di definirvi garantisti! Più che garantisti siete solo garanti della vostra parte politica a scapito dell'interesse generale del Paese. Le associazioni di volontariato che collaborano con gli enti locali e in particolare con le polizie municipali esistono già, funzionano da tantissimi anni e non hanno bisogno di questa legge. Questa legge serve solo ad autorizzare le ronde politiche per garantire alla Lega e ai pochi, fortunatamente pochi, estremisti del Popolo della Libertà il controllo del territorio. Tutto ciò aggravando i costi per i cittadini, che pagano due volte lo stesso servizio: la prima volta pagano le tasse allo Stato per avere la sicurezza; la seconda volta pagano le tasse ai sindaci per rimborsare le spese di funzionamento delle ronde. Ecco il primo grande esempio di federalismo fiscale. Speriamo che non finisca come a Padova, dove la polizia è stata costretta a scortare le ronde. Cosa dire del reato di clandestinità, una norma inutile e dannosa? perché la sanzione prevista è l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro e mi chiedo quale disgraziato che fugge dalla fame e dalla carestia, quale delinquente che viene a commettere reati in Italia si farà intimidire da un'ammenda. In realtà, questo reato non serve a nulla e le norme esistenti sulle espulsioni, sempre perfettibili, sufficienti se esistessero il personale e le risorse adeguate, che non ci sono e che non mettete. L'inefficienza dell'amministrazione non si affronta con nuove norme che, oltre ad essere eccessivamente discriminatorie, produrranno il solo effetto di intasare gli uffici del giudice di pace e di assorbire le forze residue dell'amministrazione della giustizia e degli interni in defatiganti attività, poco funzionali alla prevenzione ed alla repressione dei reati; inoltre, tutto ciò per tentare di fare qualche espulsione in più con le poche risorse messe a disposizione. l'effetto devastante di questa norma è stato profondamente sottovalutato. Essa obbligherà infatti tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio a denunciare i clandestini. La conseguenza è che che gli irregolari scompariranno d'incanto dalle statistiche, dai registri anagrafici dei Comuni, dagli ospedali, dalle scuole, dalle case e, soprattutto, dal controllo delle Forze di polizia; non scompariranno dal Paese ed alimenteranno il circuito della illegalità e della malavita. La vostra è la classica operazione di chi nasconde la polvere sotto il tappeto, ma le conseguenze di questa scelta sono drammatiche per la sicurezza degli italiani, per la reale integrazione degli extracomunitari, per i diritti della persona umana e (cosa della quale dovreste vergognarvi) per i bambini extracomunitari. Siete così accecati dal furore ideologico che ve la prendete pure con i bambini di stranieri irregolari che sono venuti o sono nati in Italia; li perseguitate, condannandoli all'apolidia, all'emarginazione e alla segregazione.

Questo provvedimento contiene inoltre delle chicche interessanti sul permesso di soggiorno a punti e sui test per i soggiornanti di lungo periodo. Avete trasformato la temporanea presenza per lavoro sul territorio in una lotteria e scambiate l'integrazione con il rispetto delle regole. Chi viene in Italia a lavorare ha il dovere di rispettare le nostre leggi; chi vuole diventare cittadino italiano, invece, non solo deve rispettare le nostre leggi, ma si deve integrare, accettando la nostra cultura, il nostro ordinamento e la nostra Costituzione. avete fatto una grande confusione: con questo provvedimento obbligate gli stranieri che vengono in Italia solo per lavorare e per periodi di tempo limitati a integrarsi, mentre gli stranieri che stanno per dieci anni nel nostro Paese e che vogliono diventare cittadini italiani non devono fare proprio nulla, non hanno bisogno di conoscere la lingua italiana, non devono conoscere e rispettare la nostra Costituzione, le nostre leggi e i nostri valori. Tutto il contrario di ciò che dovrebbe essere fatto. Questo provvedimento, signor Presidente, crea infatti solo confusione in questioni importanti per il futuro del Paese ed anche le cose buone che vi sono contenute e che noi abbiamo votato (le nuove fattispecie di reato: l'inasprimento di pena e il carcere duro per i mafiosi, l'esclusione dagli appalti per le imprese che non denunciano il racket, il sistema più efficiente per sequestri e confische, le nuove norme sullo scioglimento degli enti locali per mafia e i maggiori poteri al procuratore nazionale antimafia), rischiano di essere vanificate dalla riduzione sostanziale del personale del comparto sicurezza e, quindi, dall'eccessivo di giro di vite sulle intercettazioni che vi accingete a fare, mettendo la fiducia anche su quel provvedimento che pregiudica seriamente il contrasto, non solo alla criminalità organizzata, ma anche a quella criminalità quotidiana fatta di piccoli e grandi reati odiosi che colpiscono i ceti più deboli. Con una mano infatti introducete norme più severe e con l'altra togliete alle Forze di polizia e alla magistratura gli strumenti per reprimere i reati, anche e soprattutto quelli che voi stessi dite debbano essere perseguiti per primi. perseguiti per primi. Avete generato una grande illusione, utile forse per il breve periodo, ma dannosa per il futuro. Noi non possiamo e non dobbiamo assecondarvi; per questo diciamo no a questo provvedimento e a questo Governo.

Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, vorrei rilevare - e spero che gli italiani lo facciano con l'Italia dei Valori - che il Presidente del Consiglio chiede fiducia per il suo Esecutivo, ma si guarda bene dall'essere presente in Aula perché è evidentemente in tutt'altre faccende affaccendato. Egli stesso prova vergogna, con una maggioranza tanto ampia, a chiedere un'altra fiducia. Evidentemente è una maggioranza che non è così coesa e solida come ci volete far credere, corrosa dagli scandali che hanno investito il Premier, dal fallimento delle politiche economiche che hanno aggravato la crisi delle famiglie, dalle leggi *ad personam* approvate, come il lodo Alfano, ritornato al disonore della cronaca a causa di una cena galeotta, complici il solito Presidente del Consiglio, il Ministro della giustizia e i loro giudici costituzionali, che dovrebbero imparzialmente delibarne la costituzionalità.

intende approvare, come quella sul rientro dei capitali illecitamente esportati all'estero, un vero e proprio lavaggio del denaro sporco

che impedirà le indagini per scoprire i reati, anche quello di immigrazione clandestina e del suo sfruttamento, mettendo il bavaglio alla stampa. È un disegno di legge sulla insicurezza pubblica, per diverse grandi, enormi, insormontabili ragioni. L'Italia dei Valori aveva dato la propria disponibilità a contribuire al miglioramento del testo, con proposte emendative e ragionando con i come il Procuratore nazionale antimafia e il Governatore della Banca d'Italia, in materia di appalti e di riciclaggio. La sicurezza dei cittadini, colleghi della maggioranza, non è di destra e non è di sinistra: è un bene prezioso che dobbiamo salvaguardare, non per mero tornaconto elettorale. Voi avete seguito una strada diversa poiché l'unica sicurezza che vi interessa è quella e soltanto quella che riguarda il Presidente del Consiglio. Avete pensato bene di introdurre, fra le prime previste nel famoso pacchetto sicurezza, una norma che avrebbe bloccato tutti i processi per bloccarne uno solo, il cosiddetto processo Mills. norma ha fatto una prima comparsa per poi essere trasferita nell'aborto giuridico chiamato lodo Alfano. Poi avete aggiunto in questo provvedimento una pletora di norme manifesto, una sorta di grida manzoniana. Che dire dei medici spia e del problema sollevato dalle associazioni umanitarie a proposito dei bambini invisibili, come ricordava il collega capogruppo D'Alia? Il Governo nega però alle forze dell'ordine e alla magistratura le risorse umane, strumentali e finanziarie con cui applicare le norme, individuare i colpevoli, portarli a processo, condannarli e assicurare l'effettività della pena. Questa sarebbe sicurezza a 360 gradi, non gli *spot* elettorali

insicurezza pubblica, perché mentre si aggravano le pene per alcuni reati lo stesso Governo pone la fiducia alla Camera, e lo farà anche al Senato, sulle nuove norme in materia di intercettazioni telefoniche, norme che impediranno di indagare e di individuare i colpevoli. Ma mi rivolgo ai colleghi della Lega: ai vostri elettori lo avete detto? Nei vostri sempre più affollati comizi lo dite o non lo dite che voterete un provvedimento sulle intercettazioni telefoniche che indebolirà l'efficacia dell'azione degli organi inquirenti contro le peggiori forme di criminalità, compresa quella organizzata? Lo dite o non lo dite che state per varare una riforma della giustizia penale che anziché rendere più celeri i tempi dei processi ha sempre il solito obiettivo, e cioè salvare il Presidente del Consiglio dai suoi processi e, comunque, indebolire fortemente la pubblica accusa? E vengo al terzo motivo di insicurezza, perché il merito del provvedimento è contraddittorio. L'aver introdotto il reato di soggiorno illegale comporta automaticamente la messa fuori legge di centinaia di migliaia di persone, subito, ora. L'abnorme e irragionevole configurazione del reato è destinata a produrre una devastante azione. Altro che controllo ed efficienza del sistema sicurezza! Mettere fuori legge centinaia di migliaia di persone, renderli soggetti a sanzioni di qualunque natura li costringerà a finire nelle mani di quella malavita che li ha sfruttati e che voi, soltanto con questa norma manifesto, intendereste colpire. È una logica perversa, per cui noi riteniamo che questo provvedimento Una quarta ragione è dimostrata dalla formale abdicazione dello Stato rispetto al compito del presidio del territorio. Voi appaltate questa fondamentale funzione statale, solo e soltanto statale, a non si sa chi, né con quali poteri e con quali compiti. L'effetto di una norma del genere, come lamentato non dall'Italia dei Valori ma da tutti, dico tutti i sindacati delle Forze dell'ordine, sarà esclusivamente quello di impegnare il tempo e gli uomini della Polizia e della magistratura a dirimere e gestire le controversie generate dagli interventi dei cosiddetti volontari, in qualche caso - come dimostrano le cronache dei giorni passati - fanatici ed associazioni di fanatici che certamente non hanno alcuna competenza ed addestramento in merito. Assisteremo, quindi, ad un proliferare di rondisti in cerca di padroni politici, quando non addirittura della protezione della criminalità, o con la criminalità alle spalle per accedere ai fondi previsti. Per questo concludo ricordando non le parole di estremisti rivoluzionari, ma di associazioni cattoliche, dalle ACLI alla Caritas, dal Centro Astalli alla comunità di Sant'Egidio, dalla Fondazione Migrantes a Famiglia cristiana ed Avvenire, che ci ricordano che la sicurezza dei cittadini, delle loro famiglie, dello Stato è un bene prezioso che va perseguito con responsabilità e gestito con misura,

la forza che abbiamo nel Paese, con quella sempre maggiore che avremo e con quella che abbiamo in Parlamento. Diciamo no a questo provvedimento, no alla insicurezza per i cittadini presentata nelle forme più subdole e ripugnanti e colorata da qualche spennellata xenofoba, da fanatismo ed estremismo ma senza alcuna efficacia reale. Si dimostra, ancora una volta - e questo provvedimento ne è la cartina di tornasole - che a voi interessa salvaguardare solo e soltanto una sicurezza: quella del signor Berlusconi. La vera emergenza sicurezza, signor Presidente e colleghi, è l'emergenza sicurezza del signor Presidente del Consiglio.

con il voto di oggi su questo provvedimento, dopo aver già approvato diversi decreti-legge e ratificato accordi internazionali, completiamo il pacchetto sicurezza, voluto dal ministro Maroni e dal Governo, per rispondere alle tante e giuste richieste dei cittadini in materia di contrasto alla criminalità e all'immigrazione clandestina. In solo un anno di Governo abbiamo così mantenuto fede alle promesse fatte in campagna elettorale. In molti non lo credevano possibile, anche e soprattutto per la situazione drammatica ereditata dal Governo Prodi. È giusto ricordarlo: reati in continuo aumento, criminalità diffusa (dovuta anche all'approvazione dell'indulto), campi nomadi abusivi in ogni città, sbarchi continui di clandestini sulle nostre coste. È una riforma, quella che abbiamo realizzato, di grande responsabilità. Ci siamo arrivati dopo aver attraversato un percorso difficile, pieno di insidie, con la stampa spesso contro, con le opposizioni sempre pronte a dire no e a contestare tutto, ma con la gente e con il popolo sempre dalla nostra parte. Questa è stata, ed è, la nostra forza. Grazie a questa forza abbiamo dato il via ad una vera e propria rivoluzione politica e culturale in materia di immigrazione. Si cambia completamente rotta rispetto al passato, si abbandona per sempre il buonismo di Stato voluto dal centrosinistra, che tanti danni ha fatto a questo Paese, per portare avanti una linea di serietà e di rigore. Alla base di questi interventi legislativi c'è un concetto molto chiaro: chi entra a casa nostra lo deve fare dalla porta principale, nel rispetto della legge e, finché non ottiene la cittadinanza, rimane un ospite. Gli ospiti vanno rispettati, ma altrettanto si deve pretendere da loro. D'ora in poi, non ci sarà più posto in questo Paese per gli immigrati che non si vogliono integrare, che infrangono le nostre leggi e che vivono di criminalità, come non saranno benvenuti coloro che non rispettano la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni. *(Applausi non vuol dire rinunciare alla propria identità e alle proprie radici, come vorrebbe il centrosinistra. Integrazione, per quanto ci riguarda, vuol dire che chi viene a casa nostra (perché questa è casa nostra) deve rispettare le nostre leggi e si deve adeguare al nostro modo di vivere. Questa è l'integrazione che intendiamo noi. Abbiamo introdotto, dunque, il reato d'immigrazione clandestina. In questo modo sarà più facile e veloce espellere i tanti e troppi clandestini, che vivono non solo nell'illegalità ma anche di criminalità, di spaccio di droga, di sfruttamento della prostituzione e che si sono specializzati nei furti negli appartamenti e nelle rapine. Questa gente nelle nostre città noi non la vogliamo! Allo stesso tempo abbiamo voluto regolare la presenza degli extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno, introducendo, con un emendamento della Lega, il permesso di soggiorno a punti. Lo straniero avrà dei crediti; se non rispetta le leggi li perderà e quando questi saranno azzerati gli verrà ritirato il permesso di soggiorno e sarà espulso. Questa norma servirà per colpire quelli che non vogliono integrarsi a tutto vantaggio di quelli che, invece, si comportano onestamente. Sempre grazie a un emendamento della Lega è stata introdotta la tassa per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. Al Nord, in Padania, ma anche nel resto del Paese, la gente è stanca di pagare tasse, di pagare bolli, di pagare *ticket* e vedere che per gli extracomunitari è sempre tutto gratis e tutto dovuto. I costi dell'immigrazione devono essere anche a loro carico. Ora, finalmente, pagheranno anche loro. A questo proposito, voglio complimentarmi con i nostri sindaci, che stanno modificando le norme per le graduatorie dei servizi pubblici, assegnando ai residenti da più anni un punteggio supplementare. Gli extracomunitari sono sempre i primi nelle assegnazioni degli alloggi popolari e dei posti negli asili comunali. Questo, per quanto ci riguarda, è inaccettabile e, grazie ai nostri sindaci, anche questo finalmente finirà. Cari colleghi, noi della Lega su questi temi le idee le abbiamo molto chiare e non abbiamo paura a dirlo. Stiamo vivendo una crisi economica senza precedenti, che ha messo in ginocchio molte imprese e tante famiglie che vivono in questo Paese.

gli ultimi arrivati. Ed in questo momento, meno stranieri arrivano in cerca di un posto di lavoro meglio è. Far entrare nuovi extracomunitari vuol dire solo creare nuove sacche di disagio e nuovi disoccupati. Lo voglio dire chiaramente sia ai rappresentanti di Confindustria che ai sindacati della Triplice: il nostro Paese non ha bisogno di nuova forza-lavoro straniera. Ci sono migliaia e migliaia di nostri giovani che stanno bussando alle porte delle nostre imprese e che si sentono dire di no. Prima dobbiamo pensare ai nostri giovani ed ai nostri lavoratori; poi, come dicevo prima, agli ultimi arrivati. Questa è la realtà che evidentemente voi di sinistra, che chiedete continuamente nuovi arrivi, non riuscite a vedere. Nel frattempo dobbiamo dire grazie al ministro Maroni per il blocco dei flussi di clandestini in arrivo sulle nostre coste.

Un risultato storico ottenuto grazie anche agli accordi con la Libia e attraverso un lavoro collegiale - è giusto ricordarlo - di tutto il Governo. I respingimenti tanto contestati dal centrosinistra funzionano e nel centro di Lampedusa, che era sempre strapieno, da mesi non c'è più nemmeno un Cari colleghi, sulla linea che stiamo tenendo, noi della Lega ma anche i colleghi della maggioranza, non dobbiamo giustificazioni a nessuno. La nostra è l'unica strada percorribile per gestire il flusso migratorio in arrivo nel nostro Paese e non subire invasioni incontrollate. È giusto però rispondere alle critiche, seppur strumentali che ci vengono fatte. Chi ci accusa di razzismo si ricordi che le nuove norme che abbiamo introdotto sono già in vigore nella stragrande maggioranza dei Paesi europei, a cominciare dalla Spagna socialista di Zapatero, che negli ultimi mesi, grazie ai respingimenti - gli stessi che sta portando avanti il ministro Maroni - ha impedito a migliaia di clandestini di sbarcare sulle sue coste. Per non dire poi del reato di immigrazione clandestina, già introdotto da anni in Francia, in Germania ed in Gran Bretagna. I partiti di centrosinistra da questo punto di vista dovrebbero solo tacere anche perché, grazie alla Lega, il loro obiettivo di far entrare tutti per poi regolarizzarli, dare loro un posto di lavoro ed il diritto di voto per cercare di diventare maggioranza politica in questo Paese, è definitivamente fallito

da questo punto di vista si sono schierati apertamente dalla parte dei clandestini e contro i cittadini. Lo dimostrano ogni volta che intervengono su questi temi.

Il Partito Democratico ha impostato l'ultima campagna elettorale - lasciatemelo dire, la più vergognosa nella storia di questa Repubblica - solo sulle calunnie, sugli attacchi al Premier*,* senza mai avanzare una proposta, ma solo offese Risultato: hanno perso quattro milioni di voti. Avete perso non uno, ma quattro milioni di voti con queste vostre polemiche. La gente vi ha girato le spalle! Noi invece il consenso lo abbiamo aumentato, sicuramente anche per la coerenza e la determinazione con cui portiamo avanti le nostre battaglie, prima fra tutte quella per la sicurezza, questione che tutti i cittadini, a prescindere dall'appartenenza politica, sentono come prioritaria e sui cui si aspettano risposte da chi li rappresenta in Parlamento. risposte concrete, risposte che noi, soprattutto grazie alla tenacia ed alla visione politica del nostro segretario federale Umberto Bossi, abbiamo sempre dato, stiamo dando e continueremo a dare nell'interesse del Paese e della gente che vive sul nostro territorio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, veniamo da tre voti di fiducia richiesti per mancanza di fiducia; è una constatazione che hanno fatto anche altri colleghi, ma, insomma, occorre capire.

oltre che personale, di testimoniare un altro modo di guardare i problemi dell'immigrazione. Non voglio mettere nei guai il presidente Pisanu (ho valutato molto positivamente la sua relazione e i suoi interventi ma certo siamo in una situazione nella quale tutte le Chiese italiane, tutte le organizzazioni umanitarie internazionali, tutti i sindacati di polizia, di qualunque orientamento politico, e tutti i tecnici del settore affermano che questo provvedimento, sotto il profilo dell'efficacia del controllo dell'immigrazione clandestina, dell'assicurazione e della tutela dei beni delle persone e dell'integrità personale dei cittadini, cioè sotto il profilo della sicurezza, non funziona ed è dannoso.

è l'immagine di Marilyn Monroe, il cui volto compare pervasivamente nell'orizzonte dei *mass media* senza che tutti i consumatori dei *media* abbiamo necessariamente visto un solo film dell'attrice o ne abbiamo conosciuto la storia personale. Faccio questo esempio, ma potrei fare altri esempi di icone *pop*. *pop*. Cioè, Marilyn Monroe è di fatto svincolata da qualsiasi referente; in ultima analisi, significa solo la propria immagine. A partire da questa teoria dei simulacri, lo studioso ha poi elaborato una sua teoria della società postmoderna, vista come società dei simulacri o società simulazionale. Ecco, voi proponete all'Italia un simulacro di provvedimento sulla sicurezza, con alcune norme che significano sotto il profilo dell'immagine ma sono senza significato, direi senza senso. Che significa che una norma in un ordinamento democratico è senza senso? Significa due cose: innanzi tutto che è senza senso nell'accezione più immediata, cioè che non ha efficacia (e di questo parleremo); in secondo luogo (significato che sfugge

quindi con quel corredo di valori e di elementi del patto che tengono insieme una comunità e che vengono da essa ritenuti come indispensabile requisito di qualunque norma che abbia un senso. Voi invece introducete queste norme. Mi soffermo soltanto su quelle che sono state oggetto dei voti di fiducia, perché il resto del provvedimento è in terza lettura; mi piacerebbe mi piacerebbe che anche il presidente Gasparri si intrattenesse su queste quattro norme, che sono quelle che motivano il nostro no. In primo luogo, vi è l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, con la conseguenza di chiamata in correità di quelle famiglie nelle quali migliaia e migliaia di badanti, di colf, di *baby sitter* assicurano che ci siano bambini curati ed anziani assistiti nelle loro esigenze, che ci sia una regolarità e una serenità di vita in quelle famiglie e anche una custodia dei beni e degli averi, senza le

per migliaia e migliaia di cittadini, con l'impossibilità di denunciare la nascita di un figlio per gli immigrati irregolari sul nostro territorio, l'impossibilità di denunciare la morte di un congiunto, la negazione del diritto al matrimonio. Ciò mentre permane nel nostro ordinamento, sempre ad opera di questo Governo, il divieto dell'obbligo di non denunciare chi si rivolge a un servizio sanitario o chi, da genitore irregolarmente residente sul territorio, intende iscrivere un bambino a scuola.

né particolarmente sensibili ai princìpi e ai valori costituzionali. Ma l'aspetto che mi colpisce e che mi impressiona è che voi (l'ha detto anche qualcun altro e voglio approfondire

Voi potete anche pensare di cancellarle, potete anche costringerle a vivere nascoste. Ne parlava ieri Emma Bonino e si riferiva a una prigionia che è tale ma dignitosa,

e magari li state costringendo a consegnarsi alle organizzazioni criminali, state rischiando di creare un conflitto sociale che altrimenti potrebbe

questo Governo ha tagliato 263,5 milioni di euro per le spese della Polizia di Stato; 1,40 miliardi di euro per il triennio 2009-2011; 3,42 miliardi per lo stesso triennio a tutte le voci che riguardano la sicurezza del Paese, ossia soccorso pubblico, difesa Questo Governo prosciuga i ruoli delle forze dell'ordine perché non rimpiazza chi va in pensione. Per impiegare 3.000 militari *una tantum* sono stati stanziati 31 milioni l'anno.

dispone di 586 milioni di euro, peraltro stanziati dalla finanziaria 2008 del Governo Prodi, per il rinnovo contrattuale di 430.000 operatori delle Forze armate e della Polizia. Questa cifra basterà soltanto a coprire l'inflazione programmata per il 2009. Il 2008 è stato coperto con l'indennità di vacanza contrattuale: in altre parole, i lavoratori hanno perso un anno di aumenti che gli spettavano. Questo Governo ha tagliato sulle indennità di ordine pubblico e di missione, ma ciò non significa che ci saranno meno indagini, meno controllo e meno missioni; significa lavorare duro senza retribuzione. Gli organici calano, si impone più straordinario, ma anche quello non arriva. È incredibile - ci dica il ministro Maroni che non è così - sapere che il lavoro esterno, su strada, di un poliziotto, di una persona formata per

Allora, noi vi diciamo: piuttosto che una popolazione di invisibili, che ne direste di un lavoro serio di regolarizzazione? Il presidente Bricolo ha dovuto rivolgersi a Confindustria con parole sprezzanti, dicendo che non c'è bisogno di manodopera immigrata in questo Paese. Invece ce n'è bisogno! E un'opera di regolarizzazione

Si potrebbe proseguire sulla strada delle intese con i Paesi di provenienza, senza però avvalersi di accordi come quello tra Italia e Libia per i rimpatri illegittimi in violazione del diritto d'asilo, com'è accaduto recentemente e come recentemente ho

quello strumento, certamente l'immigrazione clandestina può essere risolta. Certamente ci vorrebbero investimenti in aiuto allo sviluppo e all'informazione. Basterebbe dire in Italia le stesse cose che diciamo quando ragioniamo del Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, che avalla la tesi secondo cui lo strumento più efficace per combattere l'immigrazione clandestina è il governo sapiente e globale dell'immigrazione regolare. gestione che costa molto meno - rifletteteci - in termini di conflitto sociale, di devianza, di forza che si attribuisce alle organizzazioni criminali, di governo della salute pubblica, di sostegno alle imprese e alle famiglie con l'accoglimento della domanda e dell'offerta di lavoro alle persone immigrate e, quindi, di sostegno al nostro sistema di *welfare* e al nostro sistema produttivo.

invita a spendere e spandere di più, diventando l'epigono di un'altra più celebre protagonista della vita del mondo che, avvertita che il popolo non aveva pane, stizzita disse: mangino *brioche*. Più o meno è quello lo spirito. Allo stesso modo voi oggi con questo provvedimento di fatto consegnate all'Italia impaurita un testo che, secondo quello che direbbe Cordero, ha la stessa identica ha la stessa identica forza di un bel pugno sbattuto sul tavolo. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, non credo di dovermi sottoporre all'esamino e alle domandine che mi sono state rivolte. Tuttavia, mentre la presidente Finocchiaro ha eluso per buona parte il merito del provvedimento, le ricordo - ed è sui banchi del nostro Gruppo un sindacalista delle forze di polizia - che il Patto per la sicurezza fatto firmare da Prodi ai sindacati di Polizia e ai COCER è rimasto lettera morta, senza una lira e senza nessuno stanziamento. Ricordo - perché lei parla di cose che conosce meno di noi, senatrice Finocchiaro, e francamente le sconsiglio di avventurarsi su questo terreno - che il Governo che lei sostenne ha lasciato le forze dell'ordine

che con l'impegno del Governo Berlusconi, del ministro Maroni, del ministro Brunetta e di tutta la nostra coalizione, è stato rinnovato il contratto 2006-2007, che voi non avete rinnovato quando eravate al Governo, lasciando senza aumenti le forze dell'ordine. sconsiglio di avventurarsi su questo terreno, perché gli argomenti sono forti e notevoli. Noi dedichiamo alle forze dell'ordine il ripristino del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che torna legge dello Stato con il voto contrario della sinistra! preferite i *no* *global* alle forze dell'ordine che nelle strade garantiscono legge ed ordine! Ora il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ritorna nell'ordinamento della Repubblica. Sull'immigrazione, voglio ricordare che il 19 giugno scorso il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri hanno ottenuto dall'Unione europea ulteriori rassicurazioni. Esiste una struttura che si chiama FRONTEX e che dovrebbe collaborare per il controllo delle frontiere e il respingimento dei clandestini. Abbiamo ottenuto impegni affinché tale struttura stanzi fondi ed aiuti l'Italia a governare questo problema. FRONTEX è passata da 80 a circa 100 milioni di euro di dotazione; ha a disposizione 25 elicotteri, 22 aerei, 24 navi, 83 motovedette ed altri mezzi. L'Italia, il nostro Governo, ha ottenuto che vengano utilizzati per respingere i clandestini che entrano

di Berlusconi, di Frattini, di Maroni e di tutto il Governo! Questi sono i fatti, nel pieno rispetto del diritto internazionale. Vede, presidente Finocchiaro, ho letto una frase su un giornale, alcuni giorni fa. Dal «Corriere della sera» del 10 maggio: se si individua con certezza il luogo da dove è partito un barcone carico di clandestini, è legittimo riportarlo indietro. Sa chi l'ha pronunciata? Piero Fassino. La differenza è che Fassino lo dice, noi lo facciamo: riportiamo i clandestini da dove partono. Non so a che mozione abbia aderito Fassino, ma mi auguro che queste posizioni trovino ascolto nel congresso del Partito Democratico, perché sarebbe una strada saggia, perdereste meno elezioni se ascoltaste queste parole, invece di fare una politica che noi non accettiamo come lezione di umanitarismo, cara presidente Finocchiaro. In questa legge si leva la patria potestà a chi manda i bambini a rubare; noi vogliamo che vadano a scuola a studiare, non a rubare! Questa è una politica umanitaria, responsabile e pedagogica, perché l'educazione è compito delle famiglie, ma anche delle istituzioni. Salutiamo quindi con grande soddisfazione questa legge, figlia di tutta la nostra maggioranza. Il Gruppo del Popolo della Libertà ha dato un contributo essenziale; condividiamo il reato di immigrazione clandestina, condividiamo tutto ciò che si fa per i centri di identificazione ed in attuazione di norme europee, che ci avrebbero consentito di fare ancora di più per trattenere i clandestini e distinguere chi ha diritto all'asilo e chi deve essere respinto. L'onorevole Fassino, giorni fa, ha affermato che è giusta la nostra politica,

di legge che contiene norme più severe sull'acquisizione della cittadinanza attraverso matrimoni, ricongiungimenti familiari e quant'altro. Per quanto riguarda le cosiddette ronde, voglio ricordare che nel provvedimento in esame si affida non soltanto ai sindaci, ma anche al prefetto (cioè ad un'autorità dello Stato) il controllo sulle associazioni volontarie, preferibilmente costituite da ex carabinieri e da ex poliziotti che aiutano a controllare le città. Meglio un ex carabiniere all'angolo di una scuola che uno spacciatore di droga

Voi fate le ronde dei delinquenti, mentre noi moltiplichiamo i cittadini onesti che controllano le città con le forze dell'ordine ed i militari!

È un pezzo essenziale del programma di Governo e oggi diventa legge dello Stato. Quindi, la questione di fiducia si giustifica perché - ripeto - abbiamo discusso per un anno, ci siamo confrontati a lungo abbiamo arricchito il testo del Governo di ulteriori capitoli; le norme antimafia sono nate dal proficuo confronto tra Parlamento (il Senato, in particolare) e Governo. Il presidente Schifani più volte nella sua posizione istituzionale aveva richiamato la necessità di un contrasto ancora più profondo alla criminalità organizzata. Ebbene, oggi approviamo questa legge che era una parte importante del patto con gli italiani. Prodi li considerava carta straccia quando incontrava le forze dell'ordine: noi rispettiamo i programmi, rispettiamo i cittadini, vogliamo più certezza della pena. Questa legge è la risposta a quelli che ci hanno

Signor Presidente, a causa di un banale incidente non ho potuto partecipare alla votazione finale del disegno di legge n. 733-B, pur avendo partecipato alle tre precedenti votazioni sulla fiducia. Naturalmente il mio voto sarebbe stato conforme a quello del mio Gruppo, in piena condivisione delle decisioni prese.

nel Consiglio energia, svoltosi a Lussemburgo il 6 giugno dello scorso anno, i Ministri europei dell'energia hanno esaminato il pacchetto legislativo sulla liberalizzazione del Mercato interno dell'energia.

oltre ai due sistemi di separazione proposti originariamente dalla Commissione, si è sviluppata una terza opzione. Originariamente si era si era pensato innanzitutto alla separazione proprietaria (nessuna società operante nella produzione, importazione o vendita di energia può avere, direttamente o indirettamente, quote di controllo in una società che gestisce reti di trasporto di energia). La seconda opzione consiste nella separazione tra proprietà e gestione, cioè una società operante nella produzione, importazione o vendita di energia può avere quote di controllo in una società che è proprietaria di reti di trasporto di energia, la gestione delle quali sia però affidata ad un'altra società totalmente indipendente dalla prima, denominata ISO *(Indipendent System Operator)*. Si è sviluppata così la cosiddetta terza opzione proposta da Francia e Germania, Paesi contrari alla separazione tra proprietà e gestione, definita ITO (*Indipendent Transmission Operator)*. Tale opzione consiste nel consentire a una impresa, verticalmente integrata nel settore energetico, di mantenere il controllo della società che gestisce le reti, ma introducendo una complessa serie di modalità operative di gestione e controllo sull'operato di quest'ultima (poteri di voto nel consiglio di amministrazione, regime di incompatibilità, monitoraggio da parte dei regolatori, obbligo di piani di potenziamento trasparenti e così via); quindi, un sistema in grado di garantire un suo funzionamento nei confronti del mercato, equivalente ad una separazione proprietaria. Ciò premesso, si fa presente che il Parlamento europeo l'11 maggio 2009 ha approvato il terzo pacchetto legislativo sulla liberalizzazione del Mercato interno dell'energia che è stato formalmente approvato il 25 giugno 2009 dal Consiglio dei ministri in seconda lettura. Nella procedura di codecisione con il Parlamento europeo è stata raggiunta la posizione di compromesso che prevede la possibilità di optare, sia nel settore dell'elettricità che in quello del gas, tra tre opzioni, come dicevamo prima: separazione proprietaria, separazione tra proprietà e gestione e *Indipendent Transmission Operator*. Al riguardo, si fa presente che al momento del recepimento di tali nuove direttive non occorrerà prevedere modifiche di rilievo della normativa nazionale vigente. In merito al secondo quesito, relativo all'indebolimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previsto da un emendamento presentato dalla maggioranza di Governo, si precisa che nella legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, non è compresa alcuna norma che indebolisce le competenze e il ruolo dell'AEEG.

Il livello decisionale europeo, tra Commissione, Consiglio dei ministri e Parlamento europeo, decisioni e codecisioni, prevede un *iter* piuttosto complesso e diverso da quello che vige nel nostro Paese.

l'ISO e l'ITO, che si differenziano in base all'operatore, integrato verticalmente oppure separato nella gestione contabile, secondo una procedura che lo stesso rappresentante del Governo definiva complessa. Mi interesserebbe sapere, quindi, e su questo dichiaro dichiaro una mia parziale soddisfazione rispetto alla risposta del Governo, qual è la posizione del Governo italiano rispetto al tema che resta sul tavolo. la posizione di monopolio, la posizione dominante dell'unico gestore distributore del nostro Paese, cioè l'ENI che, attraverso Snam Rete Gas, detiene anche la proprietà della rete di distribuzione, il mercato non si apre, non si mettono in campo manovre che favoriscono la liberalizzazione e quindi la concorrenza, a tutto vantaggio dei cittadini, degli utenti e anche della sicurezza,

sarei stato interessato ad ascoltare il parere del nostro Governo sulle opzioni che sono in campo.

Presidente, in merito all'interrogazione presentata dal senatore Stradiotto, si osserva in primo luogo che attualmente in Italia la diffusione dei punti vendita di GPL e metano, quali carburanti, è effettivamente insufficiente. Infatti, i punti vendita del GPL, sulla rete distributiva nazionale, raggiungono circa il 10 per cento e quelli per il metano solo il 3 per cento del totale. Per quanto concerne, in particolare, la rete autostradale, i punti vendita con impianti di distribuzione di gas metano in esercizio si trovano nelle Regioni Lombardia,

Circa le iniziative da assumere affinché gli enti competenti provvedano ad un potenziamento della presenza dei distributori di gas metano nella rete autostradale, si evidenzia che la normativa nazionale, recentemente modificata al fine di una più completa liberalizzazione all'accesso all'attività di distribuzione carburanti indica espressamente la promozione del miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili come, appunto, il GPL e il metano tra gli indirizzi per l'attività di programmazione del territorio delle Regioni e delle Province autonome. si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determini i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Peraltro, la modifica della normativa in materia attuata dalle Regioni sottoindicate, resasi necessaria per un adeguamento alle disposizioni nazionali e per promuovere l'uso di carburanti di minor impatto ambientale, ha condizionato le nuove autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di distribuzione carburanti. Tale modifica ha riguardato, tra l'altro, l'introduzione della prescrizione, per i nuovi impianti, dell'erogazione di almeno uno dei carburanti ecocompatibili (GPL o metano). Quanto alle ulteriori iniziative volte al potenziamento della presenza di distributori di gas metano, si evidenzia che in data 9 febbraio 2009 è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 2172, anche di mia iniziativa, recante «Disposizioni in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione». Si tratta di un'iniziativa che è stata assunta prima che io assumessi l'incarico di Sottosegretario e che, in questa nuova veste anche a nome del Governo, desidero promuovere e cercare di portare all'attenzione del Parlamento. Si fa presente, infine, che la problematica concernente la realizzazione nel futuro di una maggior diffusione dei carburanti ecocompatibili ha fatto emergere, ultimamente, una convinta attenzione anche sulle opportunità, non solo ambientali, ma anche economiche e sociali, soprattutto in riferimento al metano nel settore dei trasporti. Si fa riferimento, al riguardo, anche al recente studio realizzato da Nomisma energia che evidenzia come il valore aggiunto della filiera industriale del metano per auto può crescere entro il 2014 fino a raggiungere i 4 miliardi di euro (contro gli attuali 1,5)

ad iniziative legislative tese alla realizzazione di una rete più efficiente, più efficace e più presente di distributori di gas metano nel territorio, noi siamo ovviamente disponibili a lavorare affinché, una collaborazione tra maggioranza ed opposizione, si possa dare una risposta quanto prima a questa necessità. Tutti riconosciamo che gli autoveicoli che utilizzano GPL e metano hanno hanno un effetto positivo in termini di riduzione di emissioni di CO2, e anche dal punto di vista economico, perché permettono alle famiglie di muoversi spendendo meno rispetto ad altre fonti energetiche. quindi a disposizione e ovviamente faremo anche noi le nostre proposte per tentare di modificare quelle eventuali norme che finora hanno impedito che vi fosse la realizzazione di questi distributori.

Signora Presidente, su questo tema gli elementi di risposta sono stati condivisi con il Ministero dell'economia e delle finanze, che insieme a noi segue il tema relativo al sostegno finanziario delle piccole e medie imprese. ci sembra importante sottolineare come gli interventi di ricapitalizzazione delle banche abbiano come finalità proprio il sostegno delle imprese, dell'economia e delle famiglie. Vi è quindi, la necessità, anche attraverso un monitoraggio costante, di mantenere una relazione con gli istituti di credito, perché, accedendo agli aiuti dello Stato, possano tornare ad erogare credito in maniera sufficiente per sostenere l'economia reale. Abbiamo rafforzato il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, in particolare con un sostegno di circa 1.600 milioni di euro, che ovviamente contribuisce, in questo momento di crisi economica, a fare in modo che le piccole e medie imprese possano avere garanzie sufficienti per accedere al adottati interventi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e provvedimenti volti a favorire e accelerare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese da parte delle amministrazioni pubbliche: è annuncio proprio di questi giorni da parte del Ministro dell'economia l'intenzione di sbloccare oltre

A favore del Fondo sono stati stanziati complessivamente 1,5 miliardi di euro e a questi vanno aggiunte le risorse che, in base all'accordo quadro Associazione dovranno essere versate nel Fondo dalle banche che emetteranno specifici strumenti di patrimonializzazione, sottoscritti dallo Stato (oltre 1,5 per cento dell'ammontare degli strumenti emessi). Inoltre, è stato emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che prevede che gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, e ciò al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese alle migliori condizioni, riducendo il rischio di credito delle banche finanziatrici. In particolare, ai sensi della vigente normativa, le competenze della Cassa depositi e prestiti sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per la Cassa di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale, a 8 miliardi di euro), finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata alla concessione del credito a condizioni vantaggiose alle piccole e medie imprese. Infine, si richiamano le norme contenute nel decreto-legge n. e nel decreto-legge appena approvato dal Governo, che sono volte a favorire, anzitutto, il tempestivo pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti; poi, la riscossione di crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche anche attraverso l'intervento della SACE spa; infine, la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne le misure adottate dalla Banca europea per gli investimenti, nel precisare che l'ammontare di 30 miliardi di euro da destinare al finanziamento di piccole e medie imprese nel periodo 2009-2011 è a titolo indicativo e che non esistono quote per singoli Paesi, si fa presente quanto segue.

si è notevolmente accresciuto: nel 2008 sono stati firmati contratti di finanziamento per un importo superiore a 2,4 miliardi di euro, pari a circa due volte e mezzo l'ammontare del 2007 e quasi il 30 per cento dei finanziamenti a favore di piccole e medie imprese nell'Unione europea. Al fine di rafforzare ulteriormente questo canale di finanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze ha promosso la stipula di un accordo quadro fra Banca europea per gli investimenti, Associazione bancaria italiana e Confindustria. Questo accordo, firmato nel mese di maggio, sta già dando un nuovo impulso ai finanziamenti Banca europea per gli investimenti, anche attraverso iniziative mirate a finanziamenti attraverso banche fortemente radicate sul territorio, con una vasta clientela di piccole e medie imprese.

Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, in un momento di crisi come quello attuale dobbiamo mettere a frutto al meglio tutte le risorse disponibili per agevolare i finanziamenti al sistema delle piccole e medie imprese. Volevo semplicemente menzionare quanto contenuto nella relazione finale del governatore Draghi all'assemblea della Banca d'Italia, in cui si sottolinea la recente tendenza al rallentamento dei crediti bancari alle imprese l'indagine ISAE dell'aprile scorso che attesta un aumento del razionamento del credito nei confronti sempre delle PMI, o per rifiuto delle banche a concedere credito o perché sono le stesse imprese a rifiutare il finanziamento, perché troppo oneroso. Sono solo alcuni i dati esemplificativi per fotografare quali sono le attuali condizioni di contesto che vedono le imprese sempre più assoggettate alla stretta creditizia. Quindi tutte le misure elencate dal Sottosegretario al momento non risultano sufficienti a rispondere a questa emergenza. ai finanziamenti stanziati dalla BEI (30 miliardi di euro) da destinare ad iniziative e prestiti per le PMI in Europa nel periodo 2008-2011, non mi è sembrato sentire dalla risposta del Sottosegretario un adeguato interessamento da parte del Governo nei confronti della Banca europea per gli investimenti. Questa è una risorsa a sé rispetto a quelle che

per garantire che almeno la parte di questi finanziamenti destinati all'Italia sia cospicua e sia indirizzata proprio alle piccole e medie imprese nel più breve tempo possibile. Allo stato attuale non risultano modificate in meglio le condizioni del credito in favore delle PMI da quegli istituti cosiddetti intermediari che hanno sottoscritto contratti con la BEI per usufruire di questi finanziamenti. dovremmo riuscire a comprendere se e come effettivamente gli intermediari intendano trasmettere ai beneficiari finali, le piccole e medie imprese, i vantaggi finanziari concordati, anche in termini di tassazione agevolata; se viene rispettato l'impegno per cui ogni euro prestato dalla Banca europea per gli investimenti corrisponde a due euro di nuovi crediti alle piccole e medie imprese e se è previsto nel breve un ruolo da protagonista delle banche di credito cooperativo. Per ora nella sua relazione si è parlato soltanto di un eventuale allargamento del del ruolo di queste banche, ma ancora nei fatti non c'è. Le banche di credito cooperativo proprio per la loro presenza sul territorio possono garantire e concedere un credito alle piccole e medie imprese in maniera più semplificata e più breve rispetto al sistema creditizio tradizionale, di più ampie dimensioni, anche perché hanno un *rating* inferiore. Infine, vorrei sapere come il Governo intende verificare l'esistenza dei presupposti e quindi l'applicazione pratica delle agevolazioni stanziate dalla BEI. Non mi sembra che nella sua risposta ci sia stata una consequenzialità logica nel dire che questi finanziamenti stanziati dalla BEI vengano indirizzati direttamente a favore del sistema delle piccole e medie imprese, quindi del credito a favore delle piccole e medie imprese. Un ulteriore interrogativo che mi pongo è se questo Governo voglia facilitare accordi sul modello di quello siglato da Confindustria con ABI e BEI, al quale lei ha fatto riferimento nella sua risposta, anche per associazioni di categoria rappresentative di interessi

L'evoluzione tecnologica degli strumenti informatici resi disponibili ha portato a sviluppare un progetto per la realizzazione di uno specifico *software* per la gestione della manutenzione. Il *software* è stato realizzato ed è ora a sistema, rendendo possibile effettuare i rilievi geometrici, strutturali, conservativi, ispettivi e di valutazione della gravità degli ammaloramenti riscontrati. Già da tempo l'ANAS ha così elaborato un progetto per il rilievo e l'accatastamento delle opere d'arte e dei manufatti presenti lungo le strade statali, che si spinge fino alla determinazione dello stato di conservazione e di ammaloramento delle opere. In tal modo, ANAS si è dotata di uno strumento per la gestione della manutenzione del patrimonio stradale, mediante il quale è possibile programmare, pianificare e quantificare gli interventi di ripristino. Data l'enorme mole delle opere d'arte e degli elementi patrimoniali da accatastare e conoscere, il progetto è stato attuato dapprima per aree pilota, individuate nelle regioni Veneto, Umbria e Calabria, fino a coprire l'intero territorio nazionale. Nell'ambito delle attività di monitoraggio delle opere d'arte e dei manufatti, si inserisce il recente accordo tra ANAS e ACI, per avviare in collaborazione un programma di test sui tunnel italiani il cui obiettivo è il costante monitoraggio delle gallerie per stimolare un processo virtuoso e per migliorare gli standard di sicurezza. I test, rigorosamente indipendenti, saranno condotti da ACI senza alcuna ingerenza tra chi effettua l'indagine e il gestore del tunnel, in un'ottica di collaborazione con la commissione gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si ricorda che ANAS gestisce 1.100 gallerie, di cui 62 su rete TEN, che vanno, quindi, adeguate entro il termine prescritto indicato nel 2019, in ottemperanza alle disposizioni attuative della direttiva 54/2004 L'ANAS ha già stanziato 93 milioni di euro per un primo intervento sulle gallerie, che riguarda anche alcune gallerie della rete TEN. Per le altre gallerie è in corso un'analisi di rischio; in particolare, sono già stati avviati interventi di ammodernamento in *project financing* per un valore complessivo di 235 milioni di euro, per i 103 tunnel della rete lombarda. È un programma ponderoso, per il quale si rendono necessarie risorse imponenti, stimate in circa due miliardi di euro, per migliorare e mettere in sicurezza le gallerie, adeguandole alle caratteristiche ed ai requisiti, in termini costruttivi e impiantistici,

Attualmente, sono in corso quattro gare finalizzate ad una valutazione complessiva basata sulle analisi di rischio delle gallerie. Inoltre, gli uffici periferici dell'ANAS hanno in corso di redazione sull'intero territorio i nuovi modelli di piani di manutenzione e di piani operativi delle emergenze che verranno condivisi con le prefetture e gli enti locali interessati. Una particolare attenzione è stata dedicata dall'ANAS alle gallerie della rete stradale lombarda; è stata, infatti, stipulata di recente tra l'ANAS e la Gemmo spa la convenzione di concessione per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, un intervento che riguarda 140 chilometri La concessione, affidata attraverso lo strumento del *project financing* ed ha una durata di 21 anni (3 anni per la progettazione e 17 anni di gestione). I lavori di adeguamento tecnologico degli impianti in galleria saranno avviati entro il corrente anno e svolti senza alcuna interruzione di traffico. L'ANAS, anche a seguito dei recenti eventi sismici, ha potenziato l'impegno finalizzato ai rilievi ed alle verifiche delle opere d'arte, predisponendo i progetti e relativi servizi ai fini di prossimi appalti, per le regioni Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Lombardia importo complessivo di circa 17,2 milioni di euro), oltre a quelle già predisposte ed in fase di gara (Veneto, Umbria, Calabria per un importo di 6,7 milioni di euro). Tali aggiudicazioni avverranno entro il novembre di quest'anno. A breve seguiranno tutte le altre Regioni in funzione dei finanziamenti che saranno resi disponibili. Sono stati, altresì, predisposti, sempre per un prossimo appalto, i progetti per la regione Umbria, di prossima gara, e per la regione Campania. L'impegno totale è di circa 20,7 milioni di euro. Tutti i dati e le informazioni acquisite confluiranno nel sistema di gestione di manutenzione delle opere d'arte realizzato ed in uso presso l'ANAS.

l'aumento di traffico straordinario che vi è stato in questi cinquant'anni (va da sé che i ponti che risalgono a un secolo fa

che ricadono sotto la competenza dell'ANAS, fossero ancora in grado di assicurare gli standard di sicurezza assolutamente necessari per garantire l'incolumità di coloro che viaggiano sulle strade statali. Non solo: volevamo anche conoscere lo stato di salute dei medesimi ponti circa il possibile rischio di eventi sismici che avrebbero potuto interessare le zone in cui gli stessi ponti erano stati collocati.

parte relativa ai 5.000 ponti, che era quella più interessante e qualificante della nostra interrogazione, non abbiamo avuto risposta. Pregherei pertanto il Sottosegretario,

Nello specifico, Ferrovie dello Stato ha evidenziato le notevoli criticità emerse in relazione alla realizzazione della commessa di cui si evidenziano i principali Il progetto di ristrutturazione di 901 carrozze è stato autorizzato dal consiglio di amministrazione il 12 giugno 2002 con un costo, comprensivo di revisione prezzi e di ogni altro onere, di 282.000 per carrozza, a fronte di un programma di completamento entro il 2007. Il costo a vita intera autorizzato era pertanto pari a 254 milioni di euro. Per la realizzazione del progetto è stata esperita una gara internazionale a procedura negoziata, rivolta ai soggetti iscritti al sistema di qualificazione dei costruttori di materiale rotabile. L'appalto è stato assegnato in data 14 aprile 2003 all'unico offerente, costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese a cui partecipavano l'AnsaldoBreda (in qualità di mandataria), Firema, Keller, Ferrosud ed il consorzio Corifer. Tale raggruppamento comprendeva, di fatto, tutte le imprese iscritte al sistema di qualificazione dei costruttori di materiale rotabile, tranne due. L'aggiudicazione è stata perfezionata, con un ribasso d'asta, per un importo complessivo di 303 milioni di euro. La commessa in oggetto ha registrato, nel corso degli anni, degli scostamenti estremamente rilevanti in termini di costo e tempi, oltre ad un livello di qualità del prodotto fornito assolutamente inaccettabile. In termini di tempi, alla data del 31 dicembre 2008, erano state consegnate solo 360 carrozze, ed altre 90 erano in officina, con un ritardo quindi di oltre tre anni sul programma. In termini di costi, l'ultima stima effettuata porta il costo di 522.000 euro per carrozza, con un incremento quindi dell' 85 per cento rispetto a quanto autorizzato inizialmente. Oltre al sostanziale raddoppio dei costi e dei tempi, con l'entrata in esercizio di un consistente numero di carrozze, si sono riscontrate gravissime carenze per la climatizzazione e per le porte. In particolare, nel corso dell'estate 2008, si sono registrate delle giornate in cui il 50 per cento circa delle carrozze consegnate il sistema di climatizzazione non funzionante, con conseguenze immaginabili sulla clientela e sulla reputazione di Trenitalia. Come è noto, peraltro, i disagi per la clientela conseguenti ai citati e continui guasti all'impianto di climatizzazione di queste carrozze sono stati oggetto nei mesi scorsi anche di numerose interrogazioni parlamentari, che sottolineavano l'esigenza di individuare le cause e le responsabilità di tali disservizi. La scarsa qualità del prodotto fornito, l'allungamento dei tempi e l'esplosione dei costi hanno alterato tutto il quadro di sostenibilità economica e di attrattività del progetto, per cui, in data 13 ottobre 2008, il Consiglio d'amministrazione di Trenitalia ha autorizzato il recesso dal contratto in essere e la riduzione del numero complessivo delle carrozze da sottoporre a ristrutturazione fino ad un massimo di 450. Si evidenzia, infine, che la manutenzione dei treni Intercity citata dagli interroganti, che viene regolarmente svolta secondo le scadenze prestabilite, non ha alcuna connessione con il progetto di ristrutturazione di cui trattasi. Ferma restando la verifica del conseguimento degli obiettivi di qualità posti nel contratto di servizio con Trenitalia Spa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regolazione ad oggi in vigore e salvo quanto potrà essere statuito nell'ambito del prossimo contratto di servizio non entra nel merito degli interventi sul materiale rotabile commissionati dall'impresa ferroviaria. Eventuali profili connessi con la mancata realizzazione degli investimenti programmati possono afferire, per lo più, alle attribuzioni dell'azionista - Ministero dell'economia e finanze - ferma restando l'autonomia gestionale e decisionale normativamente attribuita alle imprese Del resto, eventuali ricadute sul piano industriale ed occupazionale esulano dalle competenze dirette del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto all'adozione di misure che effettivamente possano dare impulso allo sviluppo del trasporto ferroviario, appare effettivo e rilevante il sostegno al settore disposto

al comma 2 stanzia 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 «per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni

ringrazio il Sottosegretario per le notizie che ci ha fornito su questo problema. Prendiamo atto che ci sarebbero queste gravissime irregolarità che riguarderebbero la qualità dei materiali e i tempi di consegna. Sono notizie che ci pervengono solo ora. Noi abbiamo registrato, all'atto della presentazione di questa interrogazione insieme con il collega Viceconte nel febbraio 2009, questa situazione di ordine industriale. Una delle partecipanti al consorzio che acquisì quella commessa (la Ferrosud della Basilicata) avrebbe dovuto dar corso a una lavorazione di quasi 200 carrozze ma l'imprevista interruzione della commessa con il suo ridimensionamento da parte di Trenitalia ha determinato una condizione di crisi di questo impianto produttivo con effetti sia per i

mi permetto di avanzare un'osservazione sul sistema industriale che lavora alla costruzione del materiale rotabile, che in questi anni aveva sempre dato prova di capacità e qualità

A me non pare, onorevole Sottosegretario, di poter riscontrare nella sua risposta una rispondenza rispetto ai quesiti posti, che anche altri colleghi hanno hanno formulato al Governo. A me non pare che i difetti riscontrati o i ritardi di cui si riferisce possano giustificare un dimezzamento della commessa, da 901 a 450 carrozze. Il recesso dal contratto di cui si è parlato non ha assolutamente attinenza con tutto questo. Avrei giustificato e mi sarei spiegato un chiarimento con l'impresa e con il raggruppamento che fa capo, come soggetto mandatario, ad AnsaldoBreda. Del resto, come già affermava il collega Latronico, siamo in una condizione di crisi generalizzata dell'industria del materiale rotabile. Tale crisi si si riflette particolarmente su questa azienda, che è mandataria di questo raggruppamento temporaneo di imprese. Tale raggruppamento denota, anche attraverso un indotto che ha sede in tante unità produttive del Mezzogiorno, una qualità di servizio che fino ad oggi ha dato dimostrazione dell'esatto contrario rispetto a quanto affermato. Naturalmente non ho ragione di mettere in dubbio quanto il Governo afferma. È la risposta che non mi soddisfa; risposta che non viene posta in capo capo ai Ministeri che abbiamo interrogato (insieme ai colleghi eletti in Campania e ad alcuni altri colleghi che hanno voluto sottoscrivere la mia interrogazione). Oggi ci troviamo di fronte ad una eccellenza (che ha sede in Campania) e ad alcune altre unità produttive (che hanno sede nel Mezzogiorno) che accusano

comporteranno qualcosa come 2 milioni di ore di riduzione di lavoro presso gli stabilimenti del suddetto raggruppamento di imprese. Concludendo, onorevole Sottosegretario, a me non è chiara la valutazione dei Ministri che sono stati interrogati. Al di là delle osservazioni che adducono Ferrovie dello Stato e Trenitalia, di cui ella ha riferito, non mi pare che si possa intravedere nella risposta del Governo una intenzione di intervenire in modo tale che si possa riconsiderare la decisione del ridimensionamento della commessa di *revamping* di 901 carrozze per il trasporto passeggeri, già affidata al raggruppamento di cui è mandataria AnsaldoBreda. Né intravedo, né colgo, un atteggiamento volto ad evidenziare misure che il Governo eventualmente intendesse porre in essere per dare una mano ad un settore drammaticamente in crisi. Rispetto alla qualità del servizio apprestato fino ad oggi e dei prodotti che sono stati messi in essere nelle aziende di cui si tratta, mi sembra che fino ad oggi non si possa rilevare o eccepire alcunché. Se eccezioni ci fossero da portare avanti, sarebbe preferibile che si provvedesse direttamente presso le aziende interessate. Io credo che anche l'episodio l'episodio così duramente drammatico di Viareggio nei giorni scorsi debba insegnarci qualcosa. C'è bisogno - e concludo, signora Presidente di mettere mano ad un intervento complessivo rispetto a vetture e a carrozze che sono in uno stato di vetustà e che andrebbero restaurate o del tutto sostituite. Io credo che il Governo debba riprendere questa questione e mi auguro che lo faccia sulla base delle interrogazioni che, da più parti di questa Aula

probabilmente imporrebbe una valutazione sul metodo di capitolato, non solo nei meccanismi di rescissione.

alla paura degli immigrati di rivolgersi alle strutture sanitarie. Sulla base della legge in vigore nel settembre scorso, una ragazza ghanese di 20 anni, immigrata irregolare, è andata all'ospedale per fare un intervento abortivo ed è stata denunciata.

Orlova, una badante ucraina di 39 anni, che era incinta ed è morta dissanguata all'interno dell'appartamento in cui lavorava, a Torre a Mare, una frazione di Bari. Ha preferito prendere una bacinella e morire dissanguata piuttosto che chiamare i sanitari. Samira, un'algerina di 24 anni, ha avuto anche lei un aborto spontaneo: ha avuto una grave emorragia, non è andata all'ospedale e in questo momento è assistita dai volontari del gruppo EveryOne. Il Ministro non ha mai risposto a quell'interrogazione. Mi auguro però che il Ministro o il Vice Ministro si preoccupino di come potrebbe diventare la situazione in Italia dopo il provvedimento approvato oggi: una sanità parallela, gestita dalla criminalità organizzata, oppure una non sanità e quindi dei morti